nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011)

e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970

Sud)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, nonostante il doloroso tributo di vite umane pagato dalle Forze armate italiane per la pace e la stabilizzazione in Afghanistan e in altri critici teatri operativi, voglio ribadire che una grande Nazione come l'Italia deve rispettare gli impegni presi in ambito internazionale con le priorità e le strategie che il nostro ruolo ci impone. Il decreto va in questa direzione.

l'interesse nazionale.

un contingente di circa 9.000 militari che svolgono importanti operazioni all'estero. Con tutta la comunità internazionale contribuiamo alla stabilizzazione, alla pace, alla protezione e alla salvaguardia

e finanche al sacrificio dei nostri connazionali. Ad essi e alle loro famiglie si rivolge ancora una volta il nostro più profondo senso di riconoscenza. Lo facciamo poi anche per mezzo del personale diplomatico, di polizia e civile che, nell'ambito della collaborazione internazionale, assicura l'organizzazione degli interventi di carattere umanitario e di sostegno alle popolazioni e allo sviluppo delle economie locali. locali. Anche così si contribuisce alla pace e all'affermazione della democrazia in quelle aree del mondo. Pace e democrazia sono gli obiettivi che la comunità internazionale persegue in queste aree difficili del mondo. del mondo. È nell'ambito di questi stessi obiettivi che le operazioni dei nostri contingenti militari in ultima analisi si inseriscono. Nello svolgimento della discussione generale della scorsa settimana, anche noi abbiamo sottolineato che la decretazione d'urgenza per prorogare e rifinanziare le missioni all'estero è un pratica da superare e che si impone una vera legge in materia. Con il contributo costruttivo del Parlamento si dovrebbe varare uno strumento che assicuri un quadro normativo e finanziario stabile. Si tratta comunque di una condizione fondamentale per permettere a chi opera sul campo di pianificare e prendere decisioni nel modo migliore possibile e per impedire che all'incertezza normalmente derivante dalle operazioni in aree di crisi si sommi anche quella prodotta da un quadro normativo e finanziario incerto e potenzialmente inaffidabile. Il decreto presenta diversi punti di criticità, ivi inclusa la presenza di argomenti estranei al tema più importante. Vorrei ricordare a quest'ultimo proposito che tutti andiamo oltre il titolo dei provvedimenti che ci vengono proposti e leggiamo sempre anche tra le pieghe degli articoli. Da più parti sono stati fatti rilevare, ma riteniamo che il decreto-legge debba comunque essere convertito. È troppo importante il rifinanziamento delle missioni internazionali di pace. È un'illusione pensare che ritirando i nostri contingenti da quei territori risolveremmo i problemi. In realtà, essi andrebbero a moltiplicarsi nel tempo. Le prime a farne le spese sarebbero le popolazioni di quei territori, dove i nostri militari dovrebbero essere sostituiti da altri contingenti stranieri, con i costi legati ai passaggi di consegne e l'inevitabile incertezza in attesa che l'operatività torni a regime. Ne farebbe le spese la nostra credibilità sul piano internazionale. In un mondo che in pochi decenni è diventato piccolo, le responsabilità di un Paese come l'Italia sono automaticamente cresciute; l'impegno che abbiamo assunto nei confronti della comunità internazionale a contribuire fattivamente alla stabilizzazione, alla pace e alla democrazia in quelle aree del mondo è la diretta conseguenza di questa accresciuta responsabilità. Mostriamocene degni e difendiamo la nostra affidabilità come Paese, perché in questo momento ne abbiamo bisogno su più fronti: non solo su quello delle missioni militari, ma anche dell'economia e della politica, non dimentichiamolo.

oltre a farci venir meno a precisi impegni internazionali, creerebbe soprattutto enormi problemi ai nostri contingenti all'estero in questo particolare momento, costringendo i nostri militari a gestire una sorta di rientro in tutta fretta, probabilmente in condizioni precarie di sicurezza.

richiede tempo, e soprattutto deve scaturire da un accordo con le forze di altri Paesi in campo. Nella sua formulazione, inoltre, non tutti i Paesi hanno lo stesso peso: alcuni in particolare, per autorevolezza e presenza militare sul campo, hanno più peso. A questi ultimi, anche noi dobbiamo sottoporre al vaglio le nostre mosse, prima di una qualsiasi implementazione. la *exit strategy* non la possiamo decidere noi, qua, oggi per domani: essa va pianificata e concordata con i nostri alleati. Purtroppo, anche su questo si è fatta in questi giorni tanta inutile e controproducente propaganda, suscitando forse l'ilarità di chi ci ascolta all'estero (e accade tutti i giorni). Proprio i tristi fatti di questi giorni ci ricordano ancora una volta che per chi sta sul campo è essenziale poter contare sulla sicurezza operativa, la quale deriva in primo luogo da risorse certe e da un quadro normativo stabile per la pianificazione. Nell'auspicio che il Governo, finalmente, promuova il varo di strumenti più adeguati alla gestione di un tema così delicato, rispetto al decreto-legge d'urgenza, anche in quest'occasione non faremo mancare il nostro appoggio

signor Sottosegretario, è difficile prendere la parola oggi in quest'Aula, perché il doveroso e sentito ricordo del caporalaggiore David Tobini, ucciso in Afghanistan nel corso di un conflitto a fuoco, del quale saranno celebrati oggi i solenni funerali di Stato, coincide con il voto sul rifinanziamento delle missioni internazionali. Mi muoverò dunque su un crinale difficile per i sentimenti, ma chiaro per la ragione, riaffermando posizioni che l'Italia dei Valori ha espresso con coerenza da tempo, anche in questo ramo del Parlamento. Prima di ogni altra cosa, senza indugiare in demagogia e retorica, che nella circostanza sarebbero assolutamente fuori luogo, con vera e profonda commozione, a nome dell'intero Gruppo dell'Italia dei Valori esprimo partecipazione e cordoglio per il dolore che ha colpito la famiglia del nostro militare e il suo Corpo di appartenenza. Nell'occasione, intendo ribadire che a tutti i militari italiani impegnati all'estero in missioni difficili - le quali per l'Italia dei Valori non sono sempre compatibili con l'articolo 11 della nostra Costituzione va innanzitutto il nostro affetto per quanto fanno ogni giorno e la nostra gratitudine per il sacrificio personale, che li porta lontano dalle loro famiglie, perché essi tengono alto il nome dell'Italia fuori dai confini nazionali. Nonostante questo, proprio per quanto dirò in seguito, il no del mio Gruppo al decreto-legge in esame è sereno, ma netto e forte. «Il prezzo che stiamo pagando è altissimo per la perdita di vite umane» - in Afghanistan piangiamo la quarantunesima vittima «ma non è mai troppo alto per la sicurezza e la democrazia»; ovviamente, non sono parole mie, ma sono le espressioni del Ministro degli affari No, Ministro, la vita dei nostri ragazzi non ha prezzo, e la lotta al terrorismo internazionale - lo sa bene lei, lo sa bene quest'Aula e lo sa bene il Paese non la si può fare solo in Afghanistan, a meno che il Governo non voglia mandare i nostri soldati in ogni angolo del globo. Ancora, un altro Ministro della Repubblica «Questo è il momento del lutto, non quello di ribadire le ragioni della nostra presenza. Servono vicinanza e solidarietà». Sono le parole del ministro La Russa; ma lì, signor Ministro, non ci vanno, né i miei, né i suoi figli. Non possiamo lavarci la coscienza con il ritornello che bastano vicinanza e solidarietà, peraltro sempre fuori discussione. «Trovo incomprensibile la nostra presenza in Afghanistan e in Libia ma la Lega voterà a favore»:

afferma che «dall'Afghanistan occorre andar via. Lo dicono anche gli americani», perché obiettivo primario è «portare a casa i nostri ragazzi». Ministro e colleghi senatori, a cosa serve la nostra presenza in Afghanistan, dove siamo presenti ormai da tempo in un contesto che non è certamente oggi, e forse non lo era neppure ieri, Purtroppo, nonostante ci venga ripetuto altro, siamo percepiti, evidentemente erroneamente, come una forza di come una forza di occupazione. Sappiamo che non occupiamo quella terra lontana e che i nostri militari fanno per intero il loro dovere, ma la percezione che diamo, mettiamocelo bene nella nostra testa, ma anche nei nostri cuori, è purtroppo questa.

senza dimenticare il ridicolo balletto di Palazzo Chigi sulla Libia: prima la paura di disturbare Gheddafi, poi l'utilizzo delle nostre basi per bombardarlo, poi ancora la determinazione di combatterlo, senza dire di forniture di armi partite dall'Italia verso la Libia, di cui non si conoscono i destinatari. Per l'Italia dei Valori il nostro Paese deve rimanere leale alle alleanze e rispettare le decisioni degli organismi internazionali, ma deve essere meno interventista e più pronto alla cooperazione e alla soluzione delle questioni internazionali con ordinarie e straordinarie intese diplomatiche. La democrazia, carissimi colleghi, non si esporta mai con le armi. L'Italia dei Valori, oggi come ieri, chiede in piena coerenza una *exit strategy*, in sicurezza per i nostri militari. Dobbiamo andare via subito dall'Afghanistan, senza se e senza ma. Vorrei che la nostra presenza servisse solo per costruire strade, scuole, ospedali, e per la formazione dei funzionari della pubblica amministrazione e dei corpi di polizia interna. Ma oggi siamo chiamati in Senato a votare il decreto-legge di proroga delle missioni internazionali, che il Governo si ostina a chiamare *tout court* e sempre di pace, ma alcune delle quali restano purtroppo senza prospettive. L'Italia dei Valori dirà no al suo rifinanziamento, che costa miliardi di euro. Quando non si compra il pane in una famiglia qualche spesa va tagliata, e va tagliata subito, perché probabilmente il nostro Stato sociale è in sofferenza. È inammissibile immaginare, tra l'altro, che si continui ad assistere a questo stillicidio di vittime in Afghanistan senza fare niente. I 41 lunghissimi minuti di silenzio per ricordare le vittime sono diventati, o rischiano di diventarlo sempre di più, pura ipocrisia, anche se un'ipocrisia solenne. L'Italia deve uscire subito da questa tragica guerra, senza ulteriori, inutili e sempre deleteri tentennamenti. Vorrei ricordare che, ancora una volta, si nascondono in questo decreto-legge tutta una serie di curiosità: i balzelli e le tasse riscuotibili dalle Capitanerie di porto, le commissioni di valutazione dei vertici della Guardia di finanza, le norme per la crisi del turismo nella provincia di Trapani, le norme per favorire qualche produttore di armi. Insomma, amici, diciamolo chiaramente: in queste circostanze non possiamo nasconderci dietro il dito dell'ipocrisia.

ogni sei mesi al rifinanziamento delle missioni, apriamo una sessione straordinaria di questo Parlamento per discutere, approfondire e decidere sulle nostre missioni internazionali.

inizio col dire subito che voteremo a favore di questo provvedimento e lo faremo per due fondamentali ragioni. La prima ragione è che la partecipazione alle missioni internazionali è l'espressione più qualificante della nostra politica estera; ragione è che siamo convinti che i nostri militari impegnati all'estero meritino un sostegno incondizionato ed un'azione responsabile di tutto il Parlamento, che testimoni una comune solidarietà ai loro sforzi. In tal senso, vorrei ricordare l'ultimo tributo che il nostro Paese ha pagato per il suo impegno a difesa della pace e dell'ordine internazionale con la morte, avvenuta soltanto l'altro ieri in Afghanistan, del caporal maggiore David Tobini di 28 anni. anni. Con la fine della guerra fredda è cambiato il modo di intendere la sicurezza su scala globale, a causa dell'emergere di minacce nuove quali il terrorismo internazionale. Oggi c'è bisogno di un approccio multinazionale integrato, che risponda alle crisi non solo militari, ma anche di natura politica, diplomatica ed economica. È impossibile per l'Italia sottrarsi ad esercitare un proprio ruolo nell'ambito delle organizzazioni di cui è parte. Per questo, le Forze armate impiegate nei diversi scenari di guerra rappresentano non soltanto simbolicamente l'unità nazionale, ma sono per definizione l'espressione e l'immagine dell'Italia e sono un potente strumento di politica estera a servizio del Parlamento e del Governo. Essi sono strumento di pacificazione e di solidarietà internazionale, garantiscono la nostra presenza nel sistema delle alleanze internazionali e in organismi quali l'ONU, la NATO e l'Unione europea. Questo provvedimento tende, tra l'altro, a rimodulare il nostro impegno nella partecipazione alle operazioni di pace, prevedendo la riduzione del personale militare impegnato nelle missioni internazionali. Noi siamo un Paese responsabile; mi auguro quindi che questa non sia soltanto la volontà dell'Esecutivo, quanto piuttosto l'esigenza di corrispondere ad una ricognizione e ad una razionalizzazione rispetto al complesso delle missioni internazionali in atto, in particolare in quelle in corso da molti anni, anche da noi più volte sollecitata e rimarcata. Lo scenario afgano è quello che richiama ancora oggi maggiore attenzione. Persiste una situazione di grande instabilità, immutata dopo la morte di Osama Bin Laden. L'assassinio del fratello di Karzai, inoltre, denota la permanenza di una situazione di forte caos e confusione. La strategia di transizione messa in atto dagli Stati Uniti si sta compiendo e dovrà accompagnarsi ad un auspicabile passaggio dei poteri alle autorità locali. Questo comporta sempre maggiori investimenti a favore delle autorità indigene, ai fini del rafforzamento della loro autorevolezza e ai fini di garantire uno sviluppo socio-economico a quelle popolazioni. In tal senso, anche l'Italia è chiamata a cooperare e concorrere a questa progressiva transizione di poteri, unitamente a tutti gli altri partner internazionali, che dovrà essere graduale e dovrà assicurare sostegno alle popolazioni per un loro affrancamento e una loro progressiva una loro progressiva crescita socio-culturale ed economica. Un altro importante scenario è indubbiamente rappresentato dalla nostra sponda Sud del Mediterraneo. Penso alla crisi della Libia, ma anche alla situazione siriana. L'attuale situazione viene paragonata al crollo del Muro di Berlino, con una differenza, però, che questa volta a erigere muri è stata l'Europa. Ciò è imputabile alla lunga assenza di una politica per il Mediterraneo da parte dell'Unione europea. Risulta quindi quanto mai necessario recuperare una politica europea. Siamo di fronte ad un'occasione storica di corrispondere alle aspirazioni di tanti giovani, creando una casa comune euromediterranea, ove il rispetto delle tradizioni e delle culture sia il presupposto per costituire qualcosa di più e di diverso in nome dello sviluppo civile, sociale ed economico e dei principi della democrazia. Per questo, chiediamo con forza che il Governo diventi capofila di un piano di rinnovata politica dell'Unione europea per il bacino del Mediterraneo, che incoraggi il cambiamento dei sistemi. Non è abbandonando la Libia, come qualcuno vorrebbe far credere, che cesseranno le ondate migratorie. Solo garantendo un futuro di democrazia e libertà a queste giovani popolazioni, all'intero Maghreb e non solo e una speranza di pace a Paesi come la Somalia e l'Eritrea, che questi uomini e queste donne finiranno di rischiare la loro vita in mare. Più in generale, in tal senso appare indispensabile il reintegro dei fondi alla cooperazione allo sviluppo e alla lotta alla povertà, da sempre da questo Esecutivo penalizzate. Lo scenario africano risulta quindi particolarmente delicato. Pensiamo all'impegno nel Nord e in particolare nel Sud del Sudan, considerando la cruciale fase che ha portato all'indipendenza di quel Paese. L'impegno della comunità internazionale nelle aree di crisi africane risulta indispensabile anche nell'ottica di contrastare ogni minaccia terroristica che proviene da quelle realtà. In tal senso si colloca la nostra partecipazione alle operazioni militari di contrasto alla pirateria al largo delle coste della Somalia. Nonostante l'impegno di robusti dispositivi navali, la pirateria marittima si è diffusa in un'area di dimensioni sempre più vaste, che giunge a lambire a sud le Seychelles e a est l'India. Il provvedimento all'esame incontra quindi il nostro consenso, giacché si propone di dare concreta attuazione all'impegno contenuto nella risoluzione approvata dalla Commissione difesa del Senato lo scorso 22 giugno. Il predetto atto di indirizzo, infatti, impegnava il Governo ad individuare urgentemente soluzioni legislative in grado di superare le problematiche giuridiche connesse alla creazione di un'efficace strategia di autodifesa dei battelli civili oggetto di attacco ed a predisporre una disciplina in grado di configurare sia la possibilità di impiego di *team* armati della Marina militare, sia la possibilità per l'armatore di avvalersi di servizi di sicurezza privata a bordo delle proprie imbarcazioni. A tale proposito, voglio ricordare che nelle mani dei pirati ci sono ancora navi italiane su cui sono imbarcati marittimi italiani. È necessario quindi fare tutto quanto è nella nostra facoltà affinché i marittimi, ostaggio per atti di pirateria, possano tornare a riabbracciare al più presto i loro familiari. Prorogare la partecipazione italiana alle missioni internazionali vuol dire confermare il nostro impegno in favore di tanti processi a sostegno della pace in regioni straziate da guerre e atti di terrorismo, che coinvolgono, purtroppo, vittime innocenti. Per queste ragioni, onorevole Presidente, vogliamo ancora una volta, coerentemente, confermare il nostro sostegno a tutte queste iniziative che ci vedono ad oggi impegnati. Un impegno che, su tutti i teatri, dovrà essere indirizzato al consolidamento delle locali istituzioni e garantito fino al raggiungimento di una loro autonomia totale. Tuttavia, non possiamo esimerci dal rilevare come il sistema di finanziamento delle missioni internazionali abbia perso quei caratteri di stabilità e certezza che invece sono essenziali ai fini di garantire una seria programmazione e una serenità nella gestione delle risorse. Ci ritroviamo infatti ogni sei mesi a occuparci del finanziamento delle missioni all'estero. Dovremmo, quindi, procedere in tempi rapidi all'approvazione di una legge quadro sulle missioni internazionali che dissipi questa situazione di incertezza e non ci costringa semestralmente a doverci occupare del rifinanziamento. La ricostituzione di un finanziamento stabile, ad esempio un fondo missioni, consentirebbe inoltre di concentrare il dibattito parlamentare sulle opzioni di politica estera e di difesa. Ovvio che ciò presuppone da parte del Governo una capacità di reperire risorse stabili e concrete e un disegno politico dell'Esecutivo unanimemente condiviso e non estemporaneo, condizioni che non sempre questo Governo è riuscito a garantire; e difficilmente riuscirà a farlo da qui in avanti. Chiediamo certezze, in quanto l'incertezza di prospettive lede la dignità dei tanti uomini e delle tante donne che hanno dato e continuano a dare tanto per il nostro Paese e per la sua immagine nel mondo e mette in discussione l'operatività dello strumento militare e sua capacità di contribuire alle iniziative dell'Italia

soldati - da parte del nostro Gruppo un voto positivo su questo provvedimento. Signora Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, la Lega lo chiedeva da tempo, a Pontida lo abbiamo ufficializzato in Consiglio dei ministri i nostri rappresentanti nell'Esecutivo lo hanno fatto recepire al Governo: il «decreto missioni» che ha preso corpo per il nuovo rifinanziamento semestrale ha inserito, in maniera chiara e graduale, il ridimensionamento degli uomini nei contingenti e un abbassamento della spesa economica. La riduzione auspicata, come provano in particolare il comma 19 dell'articolo 4 del decreto-legge, che fissa al 30 settembre la data limite delle operazioni italiane in Libia, e l'articolo 9 concernente la riduzione degli organici impegnati, che caleranno di 2070 unità

È noto come la Lega non abbia condiviso fino in fondo la decisione di partecipare alla campagna promossa dal presidente francese Sarkozy, soprattutto per rovesciare il regime del colonnello Gheddafi. L'abbiamo apertamente contestata e avremmo preferito vedere il nostro Paese allineato sulle posizioni più prudenti della Germania. A questo proposito, ci pare di poter rilevare come le difficoltà incontrate finora, a quattro mesi dall'inizio delle operazioni, stiano dando pienamente ragione ai nostri dubbi di allora. Tripoli non è caduta, una sanguinosa battaglia infiamma la Sirte e le coste che erano per noi sicure non lo sono più e arriva un flusso continuo di migranti, che oltretutto i nostri *partner* europei - dobbiamo ammetterlo - non hanno nessuna intenzione di accogliere, lasciando il peso di tutto questo sulle spalle del nostro Paese. Riteniamo che i bombardamenti in Libia debbano cessare al più presto.

UNIFIL II ci ha sempre lasciato piuttosto freddi, in ragione del fatto che sin dall'inizio ritenevamo che i caschi blu non avessero i mezzi necessari a disarmare Hezbollah, come si sarebbe dovuto fare assolutamente per rendere più sicuro il Libano.

È diventato evidente che al crescere dei morti non corrispondono assolutamente dei passi in avanti compiuti dal Governo Karzai sulla strada della democratizzazione di questo sfortunato Paese. L'Afghanistan richiede un ragionamento serio, concreto, e la messa in atto di una *exit strategy*. Adesso, come tutti possono constatare, le nostre perplessità sono divenute anche quelle dell'America del presidente Obama, che proprio la scorsa settimana

Siamo convinti che presto, già dai prossimi mesi e cioè all'inizio del 2012, anche il nostro Governo trarrà dagli sviluppi in atto a livello internazionale le più ovvie conseguenze, evitando soprattutto che i nostri soldati restino soli ed ultimi a presidiare la fetta di Afghanistan loro affidata.

ad altre poste di bilancio, in particolare attingendo ben 134 milioni di euro ai fondi destinati agli interventi della Protezione civile: una cifra che non ci sembra affatto piccola. La Francia, addirittura, secondo fonti giornalistiche transalpine, avrebbe speso, nel contesto delle stesse operazioni contro Tripoli, solo 100 milioni di euro, ovvero il 30 per cento in meno. Noi riteniamo che un Paese come il nostro, che rivendica sempre di essere la settima potenza al mondo, non si può più permettere di fare il primo della classe nei teatri di crisi mondiali.

pagato in tutti questi anni e in tutte queste missioni sacrificando la loro vita. Una vita umana non ha prezzo, soprattutto se giovane come quelle donate dai nostri ragazzi adempiendo al senso del dovere. Ci sarà tempo per chiarire. Per ora ci accontentiamo dell'inversione di tendenza e del riconoscimento implicito del valore delle nostre posizioni: la diminuzione degli uomini nei contingenti e di conseguenza un minor finanziamento alle missioni,

noi riteniamo che non sia un comportamento corretto, e pertanto la Lega continuerà assolutamente sulla strada intrapresa.

numerose sensibilità, che è attraversato dal bisogno di esprimere coerentemente il proprio anelito verso la costruzione della pace

alle altre forze politiche, rispettandone, per quanto ci è consentito fare, le determinazioni assunte. Pertanto questa dichiarazione di voto, signora Presidente, colleghi, più che la manifestazione di una volontà, declinata magari all'interno di una discussione e di un dibattito talmente "domestico" da rischiare di essere dibattito "da cortile", vorrebbe poter essere un invito ad una comune riflessione e ad una condivisa assunzione di responsabilità. Presidente, colleghi, è uno dei rari momenti - benché il chiasso che mi accompagna non lo testimoni

Dovrebbe essere uno di quei momenti al limite della sacralità, nei quali tutto l'affetto e la partecipazione, tutto il sentimento - certamente onesto che noi manifestiamo nei confronti di nostri soldati quando muoiono, possa essere espresso, esternato nei confronti dei nostri soldati quando lavorano. E non può essere ritenuto da alcuno che le modalità attraverso le quali si esprime la volontà del Parlamento - quindi le condizioni in cui il lavoro degli oltre 9.000 soldati si manifesta - non siano intimamente legate al livello di credibilità che noi abbiamo come classe politica. Se noi ogni sei mesi ci ritroviamo in ad interrogarci, spesso in maniera capziosa, su questioni che il più delle volte hanno una dimensione assolutamente domestica e prescindono da una valutazione di scenario che possa conferire dignità, nobiltà e affidabilità alla nostra azione politica, come pretendiamo di poter essere considerati credibili, non solo dagli altri interlocutori politici nel resto del mondo, ma anche da quelle donne e quegli uomini che noi abbiamo mandato nei teatri a rappresentare il nostro Paese? Non basterà, cari colleghi, l'aver inserito un nostro emendamento all'articolo 9 del decreto nel quale si impone

quella prescrizione legislativa, se noi dovessimo essere orfani di un sentimento comune che ci metta nella condizione di stagliarci oltre le nostre individualità e, se mi è permesso, oltre la nostra aspirazione ad essere considerati «anime belle», nel momento in cui altri assumono su di loro la responsabilità di dare il via a che vengano indossate le divise e imbracciate le armi. Io credo che sia questo il vero crinale attraverso il quale si deve esprimere la volontà del Parlamento. La rissosità e le piccinerie della maggioranza e del Governo non intendiamo denunciarle ai fini di una bieca competizione elettorale. Lo facciamo, viceversa, per evidenziare il grave deficit che ciò determina a nostro carico sul piano internazionale. Noi come partito, lo dicevo poco fa, ad esportare non la democrazia di Bush ma affidabilità, responsabilità, coerenza, capacità di meritare la credibilità che invochiamo, sempre più spesso vanamente. Ecco perché il voto che ci accingiamo ad esprimere, che sarà un voto favorevole, vorremmo venisse considerato come il sofferto, meditato, ragionato ma convinto contributo che noi diamo non solo nei confronti dei militari che ci rappresentano, non solo nei confronti delle Forze armate delle quali abbiamo tutti i motivi per essere fieri. Le Forze armate sono un ambito di di straordinaria importanza del nostro Paese, e non sarebbe male se, una volta tanto, la politica cessasse di rivolgersi a queste con uno sguardo paternalistico, quasi a volerle avvolgere con la propria supponenza in una bolla dalla quale non potere, non dovere mai uscire. Non è solo per queste ragioni, signora Presidente, che noi esprimiamo il nostro voto favorevole. Lo facciamo perché ci preme costruire la credibilità dell'Italia; lo facciamo perché ci preme far sì che la politica

la cifra di un modo di contendere la realtà fatta davvero di piccinerie. Che tristezza, cari colleghi, vedere ridotta al rango di spesa, al rango di costo, al rango di onere finanziario la presenza, e quindi anche l'incolumità e la vita, di novemila persone nei teatri di guerra; che tristezza sentir dire da alcuni di noi che non dobbiamo più mantenere certi impegni nel teatro internazionale perché sono finiti i soldi; che tristezza dire che bisogna essere in qualche modo pacifici e pacifisti, quando poi si viene qua a chiedere la liberalizzazione nell'uso delle armi!

Noi lavoreremo per un mondo più giusto insieme a ciò che faremo per un'Italia più giusta, ma non saranno certamente né le supponenze intellettuali, né gli orgogli di fede, né le nuove ideologie ad impedirci di fare fino in fondo, come costruttori di pace ma anche come costruttori della buona e giusta politica, la nostra parte. finestra"). Colleghi, vi informo che è pervenuta la richiesta di una breve sospensione dei nostri lavori. Pertanto, sospendo la seduta fino alle ore 10,55. *(La seduta, sospesa

Signora Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, onorevoli colleghe e colleghi, ci apprestiamo a votare oggi il provvedimento di rifinanziamento delle missioni internazionali, un provvedimento che riteniamo estremamente importante. tutto ringraziare i relatori, la Commissione e la minoranza per il comportamento estremamente democratico e molto corretto.

Sappiamo anche di trovarci in un momento molto difficile, in cui molti hanno invocato il ripensamento del nostro ruolo alla luce degli ultimi eventi, che hanno scosso e addolorato

per questi valorosi combattenti, assumere l'atteggiamento di molti che, sulla scia delle emozioni, hanno chiesto di ritornare a casa, ma dobbiamo tutelare gli sforzi già profusi in questo campo. E riteniamo che ritirarsi adesso - repentinamente e contravvenendo agli accordi presi con gli Stati Uniti e la NATO sull'*exit strategy* del 2014 - significherebbe proprio questo: vanificare il nostro operato, irridendo l'impegno e l'abnegazione che le nostre Forze armate hanno speso credendo negli ideali della pace e nella possibilità assoluta di vincere il terrorismo. di vincere il terrorismo. E' possibile che le tragedie e i lutti di questi mesi abbiano fatto dimenticare il motivo per cui l'Italia è impegnata in Afghanistan? Forse. E' un motivo che non dobbiamo omettere però di ricordare: l'Italia resta lì, perché quel Paese è il serbatoio principale del terrorismo di matrice islamica, e portandovi l'ordine e la stabilità istituzionali intendiamo impedire il rifiorire delle condizioni che hanno favorito l'offensiva talebana. L'11 settembre non è mai abbastanza lontano, e fra pochi giorni, in settembre, saranno passati dieci anni da questa esecrabile tragedia mondiale. Soprattutto adesso, con l'uccisione di Osama Bin Laden, stiamo assistendo ad una forte recrudescenza delle ostilità, da ultimo con l'attentato che ha portato alla morte del fratello del presidente Karzai, e questa mattina con l'uccisione del sindaco

ma qui non possiamo cadere nelle trappole politiche: non è il caso. Bisogna piuttosto rafforzare e puntellare i nostri contingenti, dotare i nostri uomini di dispositivi sempre più sicuri, mantenere fermi gli standard qualitativi dei nostri equipaggiamenti. Non dimentichiamo l'intenso sforzo delle 4.200 unità impiegate sul campo afghano, di cui almeno 600, lo ricordo, operanti in qualità di addestratori, con l'obiettivo di rendere sempre più autonome ed efficaci le forze dell'ordine locali, il loro addestramento e la loro cultura. Solo quando sarà pienamente raggiunto tale obiettivo si potrà mettere in moto un processo di revisione. Verosimilmente, ciò non potrà avvenire prima del 2014; diamo, dunque, ai nostri soldati la possibilità di assolvere pienamente ai loro doveri nel rispetto della democrazia e della pace. Non esaminerò in questa sede

Ciò che mi spetta sottolineare oggi è il valore generale che l'approvazione di tale provvedimento implica, perché, lo ribadisco, è essenziale che tutti voi vi riconosciate nelle motivazioni appena menzionate che spingono l'Italia ad ingaggiare uomini e spendere risorse nei teatri più difficili. Ma un'altra considerazione si aggiunge ai ragionamenti suesposti. L'Italia deve mantenere i suoi impegni e non può deludere i suoi alleati: da un lato, i vicini europei, che aspettano l'irrimediabile ripiegarsi su se stessi degli americani;

L'Europa, infatti, deve fare i conti con la crisi del debito, ma anche con la prossimità geografica ai Paesi in cui assistiamo alla cosiddetta primavera araba. La guerra in Libia ha reso necessario un impegno multilaterale di molti Paesi. Sono da scongiurare, invece, le pericolose iniziative unilaterali, che disgregano il fronte e neutralizzano gli obiettivi iniziali. Per contro, gli Stati Uniti, ora concentrati sull'esplosione del loro debito, hanno discusso della possibilità di applicare la strategia del *surge and run,* non solo in Afghanistan ma anche in altri territori per loro militarmente gravosi. L'Italia, dunque, deve fronteggiare senza soluzione di continuità le sue responsabilità, consapevole che ciò deve implicare anche una seria politica di alleanze: è solo mediante la condivisione degli oneri che si possono ottenere risultati concreti. Da qui l'obiettivo di limitare l'impegno finanziario ma, nello stesso tempo, mantenere gli elevati standard di sicurezza, professionalità e operatività che contraddistinguono le nostre Forze armate, facendone apprezzare ovunque i prestigiosi contributi. È per questo, dunque, che rinnoviamo gli stanziamenti nel settore della cooperazione civile. Interveniamo, per citarne alcuni, in Iraq, in Libano, Myanmar, Pakistan, Sudan e Somalia. Siamo in prima linea nei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa sub-sahariana, e partecipiamo anche alle importantissime iniziative della Politica europea di sicurezza e difesa e ai processi di *peace keeping* dell'ONU, dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali. Per quanto riguarda, invece, la partecipazione alle missioni internazionali, inquadrata nei vari commi dell'articolo 4, bisogna mettere in evidenza l'importante somma autorizzata per la protezione dei civili in Libia. È un'operazione umanitaria vede perseguita in questo Paese la salvaguardia, se possibile, dei numerosi interessi economici che ci legano a doppio filo. La partecipazione dell'Italia origina direttamente dalla necessità di dare piena attuazione - lo si ricordi - alle risoluzioni 1970 e 1973 del Consiglio di sicurezza. Stiamo lavorando per rendere attivo il *memorandum* per il contrasto ai traffici di esseri umani: un passo importante nella lotta all'immigrazione, che ha creato seri problemi, come sapete, ai centri di prima accoglienza di Lampedusa. Grazie ai nostri sforzi si è potuto dar vita ad una missione NATO, nel rispetto della legalità internazionale, evitando che gli sforzi si disperdessero in decisioni unilaterali. Noi siamo molto orgogliosi di questo provvedimento. Ricordo la risoluzione sulla pirateria, discussa ed approvata all'unanimità dalla Commissione difesa, che mi onoro di presiedere; particolare l'articolo 5, che consente alle navi battenti bandiera italiana che si trovino in transito in acque internazionali a rischio di pirateria, di imbarcare, previa apposita convenzione ministeriale con gli armatori, dei nuclei militari di protezione della Marina

sullo stesso piano di Stati come la Francia o la Germania, fortificando le proprie navi mercantili senza che le stesse acquisiscano *de iure* lo *status* di navi da guerra. Inoltre, con questo provvedimento dimostriamo di accogliere pienamente gli stimoli e le indicazioni del Consiglio supremo di difesa, riunitosi il 6 luglio scorso.

Per questi motivi, mi auguro che si pervenga al più largo consenso possibile, in risposta anche alle esortazioni alla coesione più volte inviate dal nostro Presidente della Repubblica.

di portare la democrazia in questi Paesi. Per questi motivi, annuncio con molto piacere il voto favorevole del Gruppo Il Popolo della Libertà, nella sicurezza che questo è un passo avanti in un processo di democrazia vera e di sostegno umanitario.

Signora Presidente, la senatrice Bonino è all'aeroporto a ricevere la salma di David Tobini, mentre la senatrice Poretti è in missione con la Commissione presieduta dal senatore Marino. Annuncio quindi, anche a loro nome, la nostra non partecipazione al voto, non perché si sia in dissenso con la dichiarazione del senatore Scanu, né tanto meno perché si sia in dissenso con la presenza italiana nel mondo. L'alternativa alla presenza non è sicuramente il ritiro: l'alternativa a questo tipo di presenza la si può recuperare e proporre - noi lo avevamo tentato con alcuni emendamenti - attraverso un dibattito politico che affronti, uno per uno, i contesti e i mandati con i quali i nostri militari, cui naturalmente tutti siamo grati per il lavoro che svolgono quotidianamente, sono chiamati ad operare negli oltre quaranta teatri dove oggi sono. Qui si continua a cancellare il dibattito, a cancellare la politica e a cancellare la possibilità di onorare il ruolo che l'Italia può avere nel mondo, riducendo il tutto ad un decreto *omnibus* volto a finanziare la nostra presenza all'estero. Sicuramente, l'adozione delle modifiche all'articolo 9 rappresenta una novità importante, seppur non nella direzione da noi auspicata.

«Cari colleghi, vi scriviamo per attirare la vostra attenzione sull'emergenza umanitaria del Corno d'Africa, emergenza che ha ormai raggiunto dimensioni catastrofiche con la dichiarazione di carestia in alcune regioni della Somalia. A causa della combinazione di siccità e conflitti e al continuo aumento del prezzo dei beni alimentari, oltre 11 milioni di persone necessitano di interventi umanitari. Più di 2 milioni di bambini al di sotto dei 5 anni sono malnutriti: di questi, oltre mezzo milione sono a rischio di vita e necessitano di aiuti urgentissimi. ha lanciato un drammatico appello per salvare questi bambini, appello a cui noi non possiamo e non dobbiamo sottrarci. La nostra proposta è di devolvere all'UNICEF un giorno della nostra diaria (226 euro) per la realizzazione di alcuni interventi specifici salva-vita per i bambini del Corno d'Africa. Si tratta di un gesto fortemente simbolico ma al tempo stesso munito di grande, immediata efficacia pratica. Ecco infatti gli interventi concreti che l'UNICEF può effettuare tutti insieme e subito con la somma suddetta: acquisto di kit idrico-igienici per 20 famiglie; vaccinazione di 170 bambini; acquisto di 150 confezioni di Plumpynut (...)» (un nutriente per salvare i bambini malnutriti dalla morte per fame). Con ogni singola diaria è possibile realizzare tutti questi interventi. Il versamento della somma di 226 euro può essere effettuato con bonifico bancario, secondo le indicazioni

Signor Presidente, il disegno di legge licenziato dalla Camera e a noi pervenuto constava di sei articoli ed era volto a disciplinare l'impossibilità di ottenere l'attenuante del rito abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo. Senonché, nel corso dei lavori

veniva tecnicamente aggiustato anche per la parte riguardante il rito abbreviato.

assolutamente diversa dalla disciplina del rito. Cosa c'entrasse la disciplina della prova nel processo penale con il rito questione da noi sollevata ai fini dell'ammissibilità degli emendamenti. Il Presidente della Commissione, con valutazione

che si sono volute introdurre in materia di prova nel processo penale impattano decisamente con l'articolo 111 della Costituzione, ossia con il principio, principio, voluto dal legislatore, della ragionevole durata del processo. Si propone una modifica dell'articolo 190, comma 1, del codice di procedura penale, che attualmente è estremamente laconico

con l'articolo 111 della Costituzione, che ha introdotto il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, e con l'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della parità

Ma cosa vuol significare una cosa del genere, se non introdurre un evidente discrimine tra le parti? Ma cosa mai si è voluto dire con questa aggiunta rispetto al principio generale secondo cui le prove

una previsione di contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, ossia con la parità delle parti nell'esercizio dei propri diritti.

venga ucciso con un colpo di arma da fuoco, circostanza ricostruita attraverso il sequestro dell'arma, l'accertamento che dal caricatore manca un solo colpo, il rinvenimento del bossolo

portare mille testimoni sulla seguente circostanza: quante esplosioni di arma da fuoco siano state udite. Ovviamente la prova è pertinente,

significa che si possono portare in un processo mille testimoni per dire qualcosa di superfluo e di già accertato e che, se soltanto uno dei mille testimoni indicati non viene sentito dal giudice, il processo è nullo.

una procedura nulla, perché questa è la sanzione. Una modifica così radicale e devastante può avere una sua spiegazione, che non obbedisce alla bonifica del codice, ma ad altri fini. Ma cosa c'è di ragionevole in ciò che viene proposto? Cosa c'è di costituzionalmente protetto da questa norma? In che modo viene garantito il principio della ragionevole durata, che deve essere garantito anche dalle tattiche dilatorie di qualunque parte ossia dal costringere ad ammettere e ad assumere una prova del tutto inutile solo al fine di guadagnare tempo

Quando si salderà questo principio della dilatazione del processo con quello della prescrizione accorciata voi avrete distrutto il processo penale, il diritto dei cittadini ad avere una risposta di giustizia. Voi state

la possibilità di sentire tutti testimoni che furono utilizzati per scrivere la sentenza divenuta definitiva. Ciò va contro il principio della ragionevole durata con tante grazie della mafia, che questo vuole: e voi la accontentate.

vorrei fare una premessa, che riguarda innanzitutto il contesto di legislazione in cui si viene ad inserire la modifica che la maggioranza si accinge ad approvare. Partiamo da lontano, dalla depenalizzazione del falso in bilancio, che risale al 2002, per arrivare al cosiddetto lodo Schifani, la legge n. 140 del 2003, che è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza del gennaio 2004.

che entrano in una fascia punita da cinque a 10 anni di reclusione: guarda caso, reati contro la pubblica amministrazione, la corruzione e di criminalità economica! Si passa poi, seguendo questo breve *excursus*, al lodo Alfano, entrato in vigore nel luglio del 2008, la legge n. 124 del 2008, che il 7 ottobre 2009 fu giudicata incostituzionale dalla Corte costituzionale per violazione degli articoli 3 e 138 della Costituzione. Arriviamo così alla legge sul legittimo impedimento, la legge 7 aprile 2010, n. 51, la quale è stata dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale della Repubblica italiana nel gennaio 2011 e poi è stata abrogata per tutta la restante parte rimasta in vigore col *referendum* del giugno 2011. Ebbene, quello che si sta facendo attraverso il tentativo di introdurre il cosiddetto processo lungo finisce col contraddire sostanzialmente anche quella che è stata la volontà specifica del popolo italiano di rifiutare, attraverso il *referendum*, le norme *ad personam*. E quello che si sta mettendo in piedi altro non è che una legge *ad personam*, che presenta, come abbiamo espresso nella nostra questione pregiudiziale, dei problemi di incostituzionalità notevoli. Innanzitutto, siamo partiti da un disegno di legge che si preoccupava di evitare la possibilità di ricorso al giudizio abbreviato, e quindi ad una riduzione di pena, per i reati più gravi, quelli puniti con l'ergastolo.

non essere ammessi al rito abbreviato, con effetti devastanti sulla collaborazione alla giustizia ed il contrasto alla mafia, si giunge all'introduzione di due emendamenti, ed in particolare l'1.0.1 del senatore Mugnai, assolutamente eccentrici. Su questo punto, come ricordava il senatore Li Gotti, abbiamo chiesto una pronunzia specifica della Commissione, che stranamente si è pronunziata a favore dell'ammissibilità, malgrado l'assoluta improponibilità per estraneità alla materia ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento del Senato. Detto questo, le misure che si vogliono introdurre servono a dilatare in maniera incredibile la durata dei processi, in pieno contrasto con quello che il Governo e la maggioranza hanno fatto fino a questo momento, sostenendo il cosiddetto processo breve o - per meglio dire - il processo morto, nonché la riduzione della prescrizione prevista dalla Cirielli, facendola diventare brevissima per gli incensurati. Che cosa si fa? Si prevede una modifica al regime della prova, *ex* articolo 190, estraendo questa disposizione dalla normativa contenuta nel disegno di legge n. 1140 di riforma del codice di procedura penale in discussione dinanzi alla Commissione del Senato, e si prevede quindi che il giudice non possa più, se non a pena di nullità, espungere le liste testi, e quindi tutti i testimoni che siano assolutamente e praticamente ininfluenti. Il criterio di pertinenza e di influenza

invece, secondo questa disposizione che si vuole introdurre, la difesa ha il diritto di far sentire 30.000 testimoni, tutti gli spettatori presenti, perché sono pertinenti rispetto al fatto per cui si procede. È palese quindi la violazione dell'articolo 111, ma è palese anche la violazione degli articoli 3 e 101, poiché si sottrae al giudice la discrezionalità - per tenere il processo nei termini di ragionevole durata - di intervenire sulle liste testi e di espungere i testi assolutamente ininfluenti. Chiaramente, tutto questo produrrà l'effetto opposto; d'altronde, questo Governo e questa maggioranza per la giustizia penale nulla hanno fatto e nulla vogliono fare. Anzi, vogliono aggravare la situazione che si sta verificando, a tutto danno dei cittadini, i quali sono uguali di fronte alla legge secondo Costituzione, ma non lo sono nell'attuale situazione, in cui la giustizia penale è assolutamente inefficiente. Detto questo, la norma è aggravata dalla modifica dell'articolo 238-*bis* del codice di proceduta

Anche questa disposizione era contenuta nell'Atto Senato n. 1440, e non si capisce il motivo per cui venga anticipata in un disegno di legge che dovrebbe riguardare il giudizio abbreviato. Anche qui, la possibilità di ripercorrere tutte le dichiarazioni e tutte le testimonianze, anche se non hanno carattere di novità, significa rimettere in discussione tutta l'istruttoria dibattimentale, che magari è stata già fatta. E il caso vuole che queste due norme che si vogliono inserire siano perfettamente funzionali al processo Mills, nel quale è coinvolto il Presidente del Consiglio, da cui qualche giorno fa sono stati espunti testi dalla lista testi da parte dei giudici, e dove la sentenza passata in giudicato nei confronti di Mills fare stato del fatto storico nei confronti di Berlusconi. È evidente che noi violiamo non soltanto i princìpi costituzionali, non soltanto la Carta di Nizza, ma anche tutte le direttive europee e lo facciamo in barba ai principi costituzionali già espressi dalla Consulta. Noi abbiamo l'obbligo di celebrare i processi, e di farli celebrare in tempi rapidi, e abbiamo l'obbligo di assicurare effettivamente la parità dei cittadini di fronte alla legge. Invece, da una

dall'altro mettendo in discussione le sentenze passate in giudicato, questo provvedimento crea l'instabilità totale del sistema penale. Praticamente, la sicurezza dei cittadini va a farsi benedire, e l'unico effetto che otterremo è che salveremo una persona in danno di tutte quante le altre persone. Questa è veramente una violazione del principio di uguaglianza. Questo non significa, anche da parte del Ministro della giustizia, mettere a disposizione della magistratura, ai sensi dell'articolo 110 della Costituzione, tutti gli strumenti indispensabili perché i processi si possano celebrare. Quindi, questa norma, se possibile, è più devastante di quanto non sia la norma sulla prescrizione brevissima, perché mette in forse i processi comuni a tutti i soggetti e mette in difficoltà le parti offese: sia le parti offese, comuni sia lo Stato. Inoltre, mette in discussione i processi di mafia e si risolve in un vero e proprio regalo nei confronti della mafia, quella mafia che tutti dovremmo combattere trasversalmente: attraverso il sistema dei testimoni che possono essere riascoltati, dei collaboratori di giustizia che si possono sentire più volte, delle sentenze messe in discussione, infatti, tra poco metteremo in discussione l'esistenza stessa di Cosa nostra. Per tutti questi motivi, signor Presidente, questa normativa è profondamente incostituzionale, e come tale noi chiediamo che non possa neanche passare al vaglio del Senato e, quindi, chiediamo di non procedere all'esame del disegno di legge n.

Siamo alle solite, perché ci troviamo ad esaminare in questa Aula un provvedimento che modifica in profondità il regime di acquisizione delle prove nel dibattimento penale, a tal punto da stravolgere non solo il processo penale ma anche, e soprattutto, la disciplina costituzionale che lo regola. Si tratta, in verità, di una norma che è stata estrapolata dall'articolo 4 dell'Atto ossia una norma della riforma del processo penale che nel marzo del 2009 fu presentata dal ministro Alfano e abbandonata al suo destino in Commissione.

riguarda i poteri della Presidenza del Senato e che incide sull'*iter* di formazione della legge, sul procedimento legislativo.

soprattutto con riferimento a provvedimenti che partono in un determinato modo, che hanno uno specifico contenuto, che usufruiscono di un determinato percorso attinente all'oggetto del provvedimento stesso e poi arrivano alla fine totalmente stravolti, in violazione non solo delle regole costituzionali costituzionali che presiedono alla formazione della legge, ma anche di quel principio fondamentale che riposa nella sovranità popolare e che ha ha come presupposto la trasparenza del rapporto tra il cittadino elettore e il legislatore. Ebbene, questo è un altro esempio, un altro lampante esempio di come si viola il principio della sovranità popolare e le regole del procedimento legislativo. La Commissione giustizia del Senato aveva già incardinato l'Atto Senato n. 2567, il cui oggetto esclusivo riguardava la inapplicabilità del rito speciale di cui all'articolo 438 del codice di procedura penale ai delitti più gravi, puniti con l'ergastolo, ad esempio l'omicidio volontario. Un grande cavallo di battaglia della Lega,

quindi riguardare solo ed esclusivamente le modalità attraverso cui si escludeva dall'ammissione al rito abbreviato le più gravi ipotesi di reato, che manifestano un particolare disvalore sociale. come sempre avviene con questa maggioranza e con questo Governo, il provvedimento è stato totalmente cambiato in Commissione, ne è stata stravolto l'oggetto, il contenuto ed anche la rappresentazione per così

per oggetto, per materia, per finalità e quant'altro, fermo restando una piccola correzione, importante dal punto di vista processuale, sulla questione dei delitti punibili

perché si tratta di un provvedimento totalmente diverso da quello che è stato incardinato e proposto. Questo avrebbe consentito anche anche una maggiore serenità nell'affrontare questioni che hanno un rilievo per l'opinione pubblica di gran lunga superiore a quanto ciascuno di noi immagina.

Questa credo sia la prima delle ragioni che ci inducono a ritenere che sia necessario - non opportuno, ma necessario - non esaminare il testo che ci avete sottoposto. Quanto al merito, per brevità

rafforzare il diritto di difesa e quindi attuare quello che viene definito il principio di parità tra l'accusa e la difesa, tra le parti nel giudizio penale, meglio specificato all'articolo 111 della Costituzione, in realtà introduce uno squilibrio profondo e sostanziale. riesce a produrre, dal punto di vista normativo e concreto, una serie di effetti che sono l'esatto opposto di ciò per cui, a parole, lo si intende proporre a cominciare dalla circostanza che

mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità (...). La legge ne assicura la ragionevole durata». È evidente innanzi tutto che la condizione di parità tra le parti del processo non si realizza più, considerato che le vittime dei reati - che sono parte necessaria del giudizio penale - sono sostanzialmente pretermesse.

Il vero *dominus* del processo non è più il giudice (e, quindi, viene meno la sua funzione di terzietà), ma il vero *dominus* è l'imputato, anche per l'introduzione di una serie di sanzioni, come la nullità degli atti che riguardino l'eventuale non ammissione delle testimonianze indicate dall'imputato.

facendo l'elenco di tutte le questioni che ci riguardano. È certo, però, che ciò incide sui princìpi costituzionali, così come incide sui princìpi costituzionali la forte limitazione del potere di revoca

una violazione delle disposizioni costituzionali, e in particolare del combinato disposto degli articoli 24, 97 e 111 della Costituzione, oltre che della normativa comunitaria e di quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

norma introduce come limite e come discrimine la chiusura del dibattimento di primo grado. Ecco, ci troviamo di fronte ad un complesso di norme che dal punto di vista procedurale e sostanziale sono assolutamente in contrasto con la Costituzione. perché poi avremo altre possibilità per dare il nostro giudizio di carattere più squisitamente politico e di merito su un testo che introduce una sola cosa: l'ennesima recidiva di questa maggioranza e di questo Governo che, in violazione di ogni regola costituzionale, intendono andare avanti su una strada sbagliata, che non serve al Paese.

Le chiedo che, com'è avvenuto sempre negli anni passati, anche oggi venga sospesa la seduta, per consentire ai senatori che lo desiderano di partecipare alla cerimonia.

Signor Presidente, la vorrei pregare di interpellare il Presidente e, se possibile, di volerlo fare in tempo perché i senatori che lo desiderano possano partecipare alla cerimonia. La ringrazio.

che fa particolare riferimento alla richiesta al Senato di deliberare, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2567, che è quello che ci riguarda in questo momento. Ora, è noto, in premessa, che questo provvedimento, così com'era pervenuto all'esame del Senato e della Camera dei deputati e com'è stato poi trasmesso alla Commissione giustizia,

era stata anche avviata la discussione generale al nostro interno, salvo successivamente l'intervento di un emendamento del capogruppo del PdL in Commissione giustizia, il senatore Mugnai, che ha - di fatto e nella sostanza - completamente stravolto questo disegno di legge.

si osserva come praticamente tutti gli articoli (e cioè cinque su sei) siano stati soppressi, proprio su richiesta del senatore Mugnai, con l'emendamento cui facevo riferimento poco fa.

esisteva un nostro disegno di legge, a prima firma del senatore Maritati, e sottoscritto da tutti i senatori della Commissione giustizia del Partito Democratico, che faceva riferimento proprio al rito abbreviato ed ai procedimenti puniti con la pena dell'ergastolo, pur con l'aggravante riferita all'articolo 416-*bis* del codice penale, penale, cioè a quelli che riguardavano sostanzialmente la questione della grande criminalità organizzata di stampo mafioso. Quindi, c'era la nostra predisposizione a discutere del contenuto del provvedimento. Una volta

perché riguardava materie completamente diverse rispetto a quelle riportate nell'impostazione originale. Ci sono peraltro evidenti ragioni di natura politica e personalistica che hanno condotto a questo stravolgimento, e va anche detto che, per certi versi, ci fa specie che all'interno della Commissione giustizia, ma poi anche, almeno fino a questo momento, all'interno dell'Aula del Senato, non ci siano state rimostranze o contestazioni, o comunque segni di dissenso da parte dei senatori della Lega Nord. Infatti, a un testo di un disegno di legge a prima firma dell'onorevole Lussana che aveva una sua impostazione logica - ripeto, condivisibile o meno, comunque da discutere

ci preoccupa e ci sorprende ancora di più il fatto che sia stata per il momento accettata da tutti i senatori della maggioranza questa nuova impostazione, che ha una sola ed esclusiva logica: quella, ancora una volta, di venire a dare una mano per i problemi processuali dell'attuale Presidente del Consiglio dei ministri. Questo ci viene detto, in maniera lineare e semplicissima, soprattutto dalla norma finale che viene introdotta, quella transitoria, sulla base della quale le norme che dovrebbero essere approvate entrerebbero in vigore immediatamente, eccetto che per i processi per i quali sia stato dichiarato chiuso il dibattimento: ed è ovvio che tutti i processi dell'attuale Presidente del Consiglio dei ministri rientrano in tale fattispecie e quindi beneficerebbero di queste norme che vanno a suo favore. Detto questo, circa la *ratio* di tale emendamento e la *ratio* complessiva di questo disegno di legge credo debbano essere un attimo esaminati esaminati gli effetti deleteri, peraltro già accennati da tutti i colleghi che mi hanno preceduto, della proposta del senatore Mugnai. Non mi dilungo, ma voglio soltanto far rilevare la contraddizione che esiste tra l'intenzione di arrivare ad un processo penale possibilmente breve, o comunque il più breve possibile, e quello che invece sarebbe l'effetto pratico di tali norme. Si parla dappertutto, nelle Aule del Parlamento, nel Paese e nei dibattiti scientifici, della necessità di arrivare a norme che favoriscano l'economia processuale, e cioè l'abbreviazione dei termini processuali: qui invece si inserisce una norma che volutamente porterà ad un effetto estremamente contrario. Mi riferisco in particolare alla modifica dell'articolo 190 del codice di procedura penale, articolo per per il quale non si ravvisava assolutamente la necessità di una modifica. Infatti, così com'era impostato, il sistema processuale penale funzionava, nel senso che veniva, e viene tuttora, data a tutte le parti la possibilità di chiedere le prove e di chiedere delle audizioni testimoniali in contraddittorio e, molto correttamente, viene affidata al giudice (al presidente del collegio) la valutazione in ordine al fatto se queste prove abbiano

con intenti dilatori da parte dell'una o dell'altra parte processuale (ci riferiamo a tutte le parti processuali nel loro insieme), è necessario che il giudice

Cosa si viene ora a fare?

di qualsiasi parte di chiedere l'audizione in dibattimento di 10, 100, 1.000, 10.000 o anche 80.000 persone, se siamo nello stadio di San Siro. È perfino perfino ridicolo sostenere una tesi del genere; eppure si vuole introdurre una simile norma. Il giudice non potrà più intervenire: se 1.000 o 10.000 persone hanno visto

parlano di certezza della pena, di sicurezza, di abbreviare i tempi dei processi e poi, in senso contrario, si dilungano e danno la possibilità di dilatare in modo assolutamente assurdo ed inaccettabile questi tempi. Presidente, la mia richiesta specifica, come questione pregiudiziale in questo ambito, è che l'Aula del Senato deliberi di non procedere all'esame del disegno di legge, per consentire una valutazione in sede di Commissione del giudizio abbreviato e della possibilità di applicare o meno la diminuente prevista dal giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo, così come previsto inizialmente dal disegno di legge.

Signor Presidente, devo dire che in questo Senato non si finisce mai di uscire carichi di meraviglia.

di un disegno di legge, presentato dalla Lega, che rispondeva ad un'esigenza ben precisa: precisa: quella di escludere il rito abbreviato per i procedimenti in corte d'assise puniti con l'ergastolo. l'ergastolo. Per la verità, quando ho letto per la prima volta quel disegno di legge, l'ho trovato abbastanza interessante, perché in fin dei conti la Lega finalmente si preoccupava di giudicare

si prevede un premio a chi patteggia, ma il patteggiamento è subordinato alla confessione,

Quindi, la diminuzione di pena è strettamente legata al fatto che si fa risparmiare tempo alla giustizia, poiché chi patteggia

la possibilità di richiedere il rito abbreviato non all'inizio, ma al termine dell'udienza preliminare, prima della discussione.

l'imputato dopo aver esperito tutti i tentativi di essere prosciolto - vedendosi riconosciuto anche il diritto di difesa e di raccogliere attraverso il proprio difensore le prove a discarico a discarico valutate poi dal giudice - vede addirittura attribuita al giudice dell'udienza preliminare la possibilità di sollecitare d'ufficio la raccolta di alcune prove pur di arrivare al proscioglimento.

di cui alcuni raggiunti da prove serie e inconfutabili, una parte sceglieva il rito abbreviato per ottenere la riduzione della pena, gli altri invece andavano al dibattimento.

quantomeno nei reati di competenza della corte d'assise. Invece, cosa è successo? Per la verità, io stesso mi sono stupito, perché conosco

il processo di corte d'assise e i reati puniti con l'ergastolo, ed introducete norme che con quello che noi intendevamo proporre

in discussione un disegno di legge importante e delicato, ma nella fase della discussione e dell'illustrazione delle pregiudiziali la gran parte dei colleghi diserta l'Assemblea. Però oggi noto la presenza di autorevoli responsabili della maggioranza, quindi il mio auspicio - è un desidero profondo che manifesto - sarebbe di di sentirmi contrastare e di veder contestare ciò che sto per dire. Mi piacerebbe che qualcuno di loro mi spiegasse perché non è così come noi vorremmo che fosse quali sono le ragioni vere del provvedimento in discussione, che ancora una volta, per ragioni oscure ma non tanto, viene presentato all'esame del Senato per motivi del tutto diversi da quelli per cui formalmente si presenta un atto normativo. tratta di una procedura che definisco dal punto di vista politico e giuridico truffaldina: la tattica di presentare, sulla base di principi condivisi, provvedimenti che perseguono obiettivi totalmente opposti. Ricordava poco fa il collega D'Ambrosio che la Lega si è fatta carico di un disegno di legge che io e molti altri abbiamo apprezzato, tanto è vero che subito dopo la presentazione sono stato il primo firmatario di un disegno di legge che

del rito abbreviato, per le ragioni esposte dal collega D'Ambrosio, che non starò qui a ripetere, è uno strumento che si è andato via via deteriorando e che è stato utilizzato in maniera poco corretta. E quindi, noi eravamo aperti, disponibili concretamente, pronti a sorreggere un disegno di legge che ponesse dei limiti all'abuso di una concessione e di una riduzione consistente di pena per delitti gravissimi. Colleghi della maggioranza, spiegateci,

con gli obiettivi iniziali di contenere gli effetti negativi del rito abbreviato. Ci sarà pure una ragione per cui non volete discutere, per cui non volete ragionare e staccarvi da una linea che io definisco terribilmente dannosa per il Paese. Credo che questa legislatura passerà alla storia del Paese come quella che più ha violato i principi dell'ordinamento giuridico italiano e i principi e i valori della nostra Costituzione. Avete iniziato sin dai primi momenti a varare leggi che non avevano nulla a che

che non rende e non offre al cittadino che attende giustizia il servigio essenziale. Ma allora, di fronte ad uno sfascio di questo genere, badate, con tutte le deviazioni, con tutte le storture e, io dico, anche con tutti gli errori e gli abusi che nell'amministrazione della giustizia vengono commessi, avremmo dovuto fare fronte comune ed individuare punti di riforma essenziali che toccassero questo tema, cioè quello dei tempi terribilmente dilatati della giustizia, che cozzano con un principio che di recente è stato introdotto nella nostra Carta costituzionale, vale a dire quello Voi però non avete voluto ascoltare e ancora, con questo disegno di legge date prova di protervia e di arroganza del potere. Sapete benissimo che queste norme che state imponendo nel settore giustizia non solo non valgono a ridurre i tempi del processo, ma valgono a neutralizzare la possibilità per l'amministrazione

questo è un principio degno di discussione? È un principio giusto; ma che cosa significa affermare questo principio giusto e poi dire che il giudice viene escluso da ogni possibilità di decidere sulla rilevanza rilevanza e sull'utilità del mezzo di prova? È il momento cruciale, che fa parte della struttura, della funzione e del ruolo del giudicare

giustizia, ma non solo. Quando si pone mano ad una riforma? Quando si riscontra una difficoltà. Ed io ne ho sentite tante da parte vostra nei confronti della magistratura, veramente tante, dalla pazzia alla follia e alla politicizzazione, ma non ho mai registrato una lamentela o una circa il tema dell'assunzione dei mezzi di prova. Neppure il Presidente del Consiglio dei ministri, se non ricordo male, ha mai lamentato che i suoi avvocati abbiano prodotto richiesta di assunzione di mezzi di prova e questi siano stati proditoriamente non accolti. Non esiste questo problema nel Paese, e

Perché lo fate? Lo fate evidentemente per servire gli interessi di una persona, e poi nel vostro interesse, per mantenere insieme una maggioranza che vacilla. Non volete andare a casa? Va bene, lo capisco. Volete concludere questa legislatura? D'accordo, ma in uno scorcio di legislatura, vogliamo assumere un comportamento che sia almeno minimamente dignitoso verso i principi della Costituzione? Perché non variamo norme che non tocchino i problemi del Presidente del Consiglio dei ministri, ma che possano valere, sia pure in minima misura, ad agevolare l'attività giudiziaria? Con queste norme non faremo altro che paralizzare ulteriormente il funzionamento - ripeto - già asfittico, difficile e quasi impossibile dell'attività giudiziaria. Siete ricorsi ai lodi,

L'Assemblea legislativa legifera in maniera generale, prescindendo da interessi particolari. Voi ci state imponendo un'attività di legislatura che invece, al contrario, è diretta a garantire interessi privati.

Perché si possono interrogare nuovamente, riesaminare, anche sulla base di queste tecniche di intimidazione, tutti i testimoni le cui dichiarazioni sono state utilizzate per decidere e scrivere una sentenza passata in giudicato. A cosa serve questo? A sostegno di quale diritto? forse che tutti i giudici che scrivono sentenze siano sospetti? Siete tornati alla teoria della pazzia, oppure siete tornati alla teoria della pericolosità dei magistrati? Allora abbiate il coraggio di fare una riforma costituzionale che abroghi la magistratura e modifichi addirittura i principi successivi

Non abbiamo alcun interesse specifico a richiamare l'attenzione su questo punto. Abbiamo piuttosto l'interesse che deriva dal nostro ruolo di rappresentanti degli interessi collettivi. Con queste norme non serviamo gli interessi collettivi, ma li danneggiamo. Oggi c'è un deliberato del Consiglio superiore della magistratura che invito a leggere. Non lo leggo in questa sede

l'entusiasmo e la fede che ancora mi contraddistinguono questo intervento, e l'ho rivolto a voi, amici della maggioranza, nella speranza che almeno questa volta

Ci sono stati dei quesiti referendari, e l'elettorato italiano, compresa una maggioranza degli elettori del centrodestra,

Questa è una notizia, perché è come dire che è l'uomo che morde il cane, e non viceversa. Si poteva benissimo pensare che, avendo quattro schede a disposizione, coloro che hanno votato per il centrodestra alle elezioni politiche ritenessero sensata la scelta di fare leggi *ad personam*, purché il proprio Governo governasse. Però, più della metà degli elettori del centrodestra ha votato sì: un ragionamento che è un'aggravante, tanto più se si considera, come tutti noi abbiamo rilevato, che dopo l'intervento della Corte costituzionale quel testo di legge era stato sostanzialmente depotenziato,

Come è possibile allora, in termini politici, da parte di un centrodestra che si sente in difficoltà e che vuole rifondarsi, ripartire con una nuova legge *ad personam*? Questo è il problema politico serio, perché il Paese ha bisogno, per far funzionare bene la democrazia dell'alternanza, che i due poli siano entrambi fungibili, ragionevoli e che vogliano intervenire. Per cui tutti siamo interessati a che per entrambe le parti dello schieramento politico ci sia una fase di bipolarismo nuovo. Ma se voi, con la nuova legge *ad personam*, sfidate i vostri elettori, che vi hanno sfiduciato su questo punto, allora dovreste cambiare il nome della Costituente che volete fare, e non chiamarla Costituente popolare, bensì Costituente impopolare. Voi vi battete contro il vostro popolo, che vi ha sconfessato su questo. Dovreste quindi riflettere, nel vostro interesse, prima che nell'interesse del Paese, sul fatto di non ripercorrere una strada dannosa per voi, per la credibilità anche di un nuovo centrodestra che volete rifondare. non si può non fare una seconda valutazione di contesto. Ieri, alla Camera dei deputati avete votato una questione pregiudiziale di costituzionalità sull'omofobia

Ma come? Ieri alla Camera dite che il principio di uguaglianza formale va difeso in maniera così intransigente che, anche rispetto a una minoranza discriminata, si vota una pregiudiziale di costituzionalità, e oggi al Senato, viceversa, per la persona del Presidente del Consiglio, quella uguaglianza formale ieri così sacra e intangibile diventa negoziabile e derogabile, a distanza di

vale per l'omofobia, varrà un po' di più per il Presidente del Consiglio, che, rispetto ad una minoranza discriminata, mi sembra abbia un potere economico e politico ben superiore. Vengo al merito. La nostra questione pregiudiziale propone due osservazioni in premessa. riguarda il modo di fare legislazione che si verifica anche in questo caso, usando un provvedimento che passa come cavallo di Troia per riconvertirlo in uno di tutt'altra natura, e quindi questo modo estemporaneo e disorganico di fare leggi. La seconda riguarda cosa noi facciamo del quinto comma dell'articolo 111 della Costituzione, in particolare con le modifiche all'articolo 1, che finiscono per annullare i vantaggi di economia processuale del rito abbreviato.

111 che impone alla legge di regolare «i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto effetto di provata condotta illecita». Esso è un punto cardine perché, come riportano anche i commentari della Costituzione, solo se si riconduce a ragionevolezza e si ammettono talune deroghe, il metodo del contraddittorio può effettivamente essere utilizzato e rispettato.

La prima è che in maniera irragionevole viene colpito il ruolo di snodo e di filtro del giudice. Infatti, se l'imputato ha sempre diritto di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni del pubblico ministero, il ruolo del giudice è quello di chi è costretto ad ammettere anche prove superflue per obbligo di legge, tutto il ruolo di discrezionalità del giudice viene scardinato. E tanto più questo

per andare deliberatamente verso la prescrizione. L'obiettivo non è più un processo, né breve né lungo, ma un processo che, a tappe forzate, restringendo il ruolo del giudice, va verso la prescrizione. la ragionevole durata del processo, con questa riforma condivisa che abbiamo fatto dell'articolo 111 della Costituzione, va a farsi benedire. terza e ultima considerazione - c'è il problema dell'assenza di una norma transitoria di salvaguardia dei giudizi già instaurati, che rivela la natura di norme *ad personam*. In particolare, il comma 5 dell'articolo 1, limitandosi a derogare per i processi in corso alla data di entrata in vigore quando sia stata già dichiarata la chiusura del dibattimento di primo grado, vuole deliberatamente far salvi i processi per il Presidente del Consiglio dei ministri. E qui ritorniamo al punto di partenza, non solo costituzionale, ma politico, cui accennavo prima. É possibile ragionare di leggi *ad personam* dopo 15 anni, come se il vostro elettorato, e non solo il nostro, non vi avesse solennemente sconfessato? Perché qui non è in gioco solo la costituzionalità, ma anche la ragionevolezza politica, che vi dovrebbe indurre a prendere atto dei risultati di quel *referendum*, per quello che significano, al di là del voto sulla scheda gialla.